Senatore Viceconte, Signor Presidente, la mia replica sarà molto breve, per due ragioni. La prima é che in realtà l'impianto complessivo del testo che è venuto dalla Camera e del testo approvato in Commissione sostanzialmente Commissione sostanzialmente viene condiviso - salvo un aspetto di cui dirò fra un momento - dai colleghi della maggioranza e dell'opposizione, gli elementi della riforma sono stati ben illustrati sia da me che dal collega Morando e ben individuati nel dibattito. Ciò che rimane aperto sarà meglio espresso in sede di parere sugli emendamenti, perché rimangono dei dei punti sui quali l'opposizione e la maggioranza hanno al momento opinioni diverse. Essi riguardano due aspetti fondamentali: per un verso, l'introduzione in questa legge di alcuni parametri che stanno costituendo oggetto di dibattito in sede europea che a breve li introdurrà, però, direi in maniera profonda, all'interno dell'intero sistema economico dell'Unione europea; per altro verso, alcune proposte che riguardano le strutture di supporto tecnico al lavoro del Parlamento, che in questo contesto dovrebbero assumere un particolare significato. Sono questi i temi che in questo momento non trovano una condivisione da parte dei colleghi della maggioranza e dell'opposizione e che sarà meglio affrontare, ribadisco, al momento dell'espressione dei pareri sugli emendamenti. Vi è altresì una modifica approvata in Commissione e sulla quale si è discusso, ma si è rimasti anche lì di parere leggermente diverso, relativa a una migliore migliore redazione del bilancio di cassa, nel quale ritrovano un loro

più efficace il bilancio di cassa e nel contempo, attraverso gli elementi di competenza, consentono una migliore programmazione dell'intera azione economica e finanziaria dello Stato.

alle nuove esigenze della *governance* economica europea. Sappiamo quanta rilevanza ha ancora adesso questo problema; sappiamo quanto sia necessario che le politiche di rientro dal debito e le politiche finanziarie degli Stati membri dell'Unione europea e sappiamo quanto il problema della competitività sia rilevante per

è dunque assolutamente importante, direi essenziale, perché per un verso favorirà l'azione del Governo all'interno dell'Unione Europea e per altro verso altro verso marcherà la politica di rigore nei conti pubblici che il Governo ha adottato finora, ponendo, nel contempo, le premesse di tipo metodologico per un nuovo patto di competitività e crescita che si si auspica possa riportare lo sviluppo in sede europea ma anche, e soprattutto, in sede italiana. minoranza*. Signor Presidente, in questa sede e in attesa di illustrare gli emendamenti che abbiamo presentato al disegno di legge così come modificato dalla Commissione bilancio vorrei limitare le mie osservazioni a qualche giudizio sull'orientamento politico generale che emerge, per quello che riguarda la maggioranza, dal dibattito e dalla replica che ha appena tenuto il relatore. Per farlo vorrei ripartire dalla domanda che io stesso ho posto nella relazione di minoranza qualche giorno fa. Poiché quando

si presenta con la volontà e l'obiettivo di resistere alle innovazioni che verranno introdotte nella nuova *governance* e nel coordinamento delle politiche di bilancio dell'Europa cercando in quella sede, in buona sostanza, di chiedere uno sconto - in nome di elementi di forza del nostro sistema economico che sono stati più volte richiamati in questo dibattito e che sono reali - rispetto al rigore che caratterizzerà l'orientamento dei Paesi più forti in quel contesto e più rigorosi, come i Paesi dell'area del marco? Oppure l'Italia è orientata a partecipare a questo confronto sulla base di un orientamento diametralmente opposto, cioè far valere i punti di forza che caratterizzano il nostro sistema economico nel contesto europeo

concedere al nostro Paese, in nome di un'antica solidarietà, uno sconto rispetto al rigore, allora nella

che è previsto come fondamentale documento per il coordinamento delle politiche economiche e delle politiche di riforma alla dimensione europea. Insomma, se alla domanda che ho posto rispondiamo

metterci a posto sul terreno di un orientamento solido per il risanamento della finanza pubblica, in modo tale da presentarci già al Consiglio europeo del 24 e 25 marzo come un Paese consapevole della sua forza, che c'è e sfida gli altri Paesi ad un coordinamento delle politiche economiche e di bilancio coerente con le esigenze risanamento finanziario e di stabilizzazione finanziaria, ma soprattutto di crescita e di maggiore coesione sociale. Per esempio, ci presenteremmo nell'avanzare la proposta dei cosiddetti eurobond per finanziamenti infrastrutturali, sul merito di credito dell'Europa, o nel proporre che quote crescenti di debito pubblico in Europa siano gestite alla dimensione europea, sul merito di credito dell'Europa e non dei singoli Paesi (quote proporzionali alla ricchezza, al prodotto interno lordo, e non al volume globale del debito, ovviamente, di ogni Paese). Se dunque pensiamo che il nostro Paese debba presentarsi in quella sede forte degli elementi di robustezza della nostra economia, consapevole dello squilibrio macroeconomico legato al volume troppo grande del debito pubblico in Italia, e per questo orientato ad ottenere nella sede europea una svolta, un rivolgimento vero e proprio degli orientamenti di politica economica prevalsi nell'attuazione del Patto di stabilità e di crescita e nella mancata attuazione del Trattato di Lisbona nel corso di questi anni, allora è chiaro che dovremmo utilizzare l'occasione della riforma della legge di contabilità

Badate che non sto dicendo e proponendo nulla che non sia ciò che stanno decidendo le principali Nazioni. Illustrando l'emendamento che propongo a questo proposito, leggerò all'Aula (così almeno la smettiamo di dire che ci stiamo occupando di cose che riguardano il 2015, il 2016, o non si sa quando), la Germania abbia già adottato, modificando l'articolo 115 e l'articolo 109 della sua Costituzione, nella sua Costituzione Costituzione nazionale, le regole che consentono di rendere più credibile il rispetto del Patto di stabilità e di crescita.

Guardate che si tratta di un orientamento assai pericoloso. Leggerò, presentando l'emendamento (adesso voglio concludere), la parte del documento firmato da Silvio Berlusconi come Presidente del Consiglio dei ministri, al termine della riunione dell'11 marzo, documento nel quale il Presidente del Consiglio italiano si impegna ad adottare, già per il 24 e 25 marzo, misure di riforma nella legislazione nazionale che siano coerenti con il Patto di stabilità e di crescita,

che, a proposito dell'obiettivo del pareggio di bilancio, reagendo a una polemica di altri Ministri che lo accusano di non finanziare, così danneggiando, la campagna elettorale del centrodestra imminente, o in corso, amministrative per le amministrative, reagisce a queste critiche dicendo (cito

«ma poi, la firma sotto l'obiettivo del pareggio di bilancio ce l'ha messa il Presidente del Consiglio, non ce l'ho messa mica io!». Ma allora, qualcuno nel Governo lo sa, che c'è quella firma. Presentando gli emendamenti, leggeremo i testi, in maniera tale che risulti che sta accadendo in quest'Aula e nel dibattito di politica economica nazionale qualcosa di assolutamente paradossale. L'Europa sta decidendo per una svolta - come che la vogliamo giudicare, naturalmente - nel coordinamento delle politiche economiche e di bilancio. L'Italia in sede europea partecipa, debbo dire consenziente, agli orientamenti prevalenti in quella sede; dopodiché coloro che in quella sede prendono decisioni impegnative per tutti vengono in Italia e dicono che quelle decisioni non esistono. Penso che questo tipo di orientamento sia dannoso per il Paese; poi forse è dannoso anche per il centrodestra, ma degli interessi del centrodestra se ne occupa il centrodestra. Noi cercheremo di occuparci un pochettino degli interessi del Paese e di quelli del centrosinistra e, alla luce di questo banale posizionamento, pensiamo che l'occasione della legge di contabilità dovrebbe essere usata per introdurre quelle innovazioni di cui ho parlato. Ancora confido che, illustrando gli emendamenti, e poi il relatore di maggioranza e il Governo dando il parere sugli stessi, possa prevalere ciò che a questo punto è un elemento di mero buon senso e di coerenza rispetto all'orientamento che lo stesso Governo sostiene alla dimensione europea. Se non sarà così, naturalmente, nell'orientare le nostre decisioni di voto, saremo conseguenti.

parere non ostativo». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta».

l'emendamento 2.2 affronta il tema del Patto di stabilità e della possibilità di coinvolgere le Regioni nel rispetto dello stesso.

Ci sembra che questa norma vada nella direzione del federalismo di cui stiamo discutendo in questi giorni, perché consente alle Regioni di avere un ruolo molto attivo e molto importante sul Patto di stabilità.

A pagina 10 di questo documento, che tutti i senatori hanno avuto, perché è stato diligentemente distribuito dagli Uffici del Senato, sta scritto quanto leggerò (scusatemi per la pedanteria, ma la situazione è veramente paradossale). «Regole di bilancio nazionali» (questo è il titolo). «Gli Stati membri della zona euro si impegnano a recepire nella legislazione nazionale le regole di bilancio dell'UE fissate nel patto di stabilità e crescita. Gli Stati membri manterranno la facoltà di scegliere lo specifico strumento giuridico nazionale cui ricorrere ma faranno sì che abbia una natura vincolante e sostenibile sufficientemente forte (ad esempio costituzione o normativa quadro)». Sotto questo documento c'è la firma di Silvio Berlusconi.

Nel 2005, non ieri mattina, il Patto di stabilità e crescita era considerato troppo prociclico, cioè stupido, per usare l'espressione del presidente Prodi: un patto, cioè, che quando le cose vanno male le fa andare peggio, e quando vanno bene le fa andare un po' meglio. Un patto quindi assolutamente prociclico, incapace di organizzare una politica economica e di bilancio alla dimensione europea che reagisca in positivo all'andamento della crisi. Cosa si diceva

ad un obiettivo espresso in termini di indebitamento strutturale. Cosa è l'indebitamento strutturale? È l'indebitamento corretto per l'andamento del ciclo, in maniera tale che la correzione sarà molto più grande da fare, se non si è raggiunto l'obiettivo di medio termine, cioè l'obiettivo del pareggio, se le cose vanno bene, perché i margini nell'economia ci sono per un miglioramento della finanza pubblica; fermo restando che, quando nell'economia le cose andranno male, si potrà fare una politica fiscale più espansiva. Qual è l'obiettivo di medio termine dell'Italia già fissato nel Patto del 2005? È il pareggio di bilancio strutturale entro dieci anni: 2005-2015.

deve migliorare ogni anno dello 0,5 per cento rispetto all'anno precedente il dato dell'indebitamento strutturale. Quando i Capi di Governo mettono la loro firma sotto un documento che

una ridefinizione del Patto di stabilità e crescita. L'emendamento 2.4 (testo 2), se voi lo leggete per un attimo, prevede infatti che l'obiettivo di medio termine fissato nella legislazione è il pareggio di bilancio strutturale;

Questa scelta naturalmente è molto impegnativa ma non è nuova, colleghi: è semplicemente l'inserimento nelle regole della decisione di bilancio nazionale e di gestione della finanza pubblica nazionale di un'ulteriore regola già decisa. La novità è che l'Europa la renderà esigibile. Come? Con il passo che vi ho appena letto. La dimostrazione che le cose stanno così, signor Presidente, è data dal fatto che la Germania

assolutamente anticiclica, ma con deroghe fissate dalla legge e con *quorum*, addirittura, di voto del Parlamento per derogare a quegli orientamenti. Ma si dice: la Germania è la Germania, troppo forte, sta troppo bene... Ma la Francia non è affatto in condizioni di bilancio particolarmente diverse, per quello che riguarda l'indebitamento annuale, rispetto all'Italia; anzi, l'indebitamento 2010 è decisamente peggiore per la Francia di quanto non sia per l'Italia.

almeno tre anni, ma meglio cinque - sono tali da determinare come conseguenza che una legge di bilancio annuale che non rispetti lo sforzo programmato dalla legge pluriennale come definita in Costituzione sarà annullata in quanto contraria alla Costituzione. In sostanza, i francesi introducono in Costituzione una norma che stabilisce che se il Parlamento adotta una legge di bilancio annuale contro lo sforzo di coordinamento e di risanamento fissato dalla legge pluriennale come da modifica costituzionale, quella legge di bilancio dovrà essere annullata. annullata. Signor Presidente, lei sa bene quanto sia cruciale il potere di bilancio di un Parlamento: si tratta quindi di una decisione di portata veramente straordinaria. Il documento conclude: «L'iscrizione di questo testo all'ordine del giorno del Parlamento permetterà a ciascuna delle Camere

- non faremo altro che scrivere ciò che ci siamo impegnati a fare nella legge di contabilità, potendo il 24 e il 25 marzo andare in Europa a dire quello che dovevamo fare, come la Germania e come la Francia, lo abbiamo già fatto, perché il Senato ha approvato una legge che contiene queste nuove regole che abbiamo deciso, assieme, di adottare. Naturalmente, potremo ulteriormente sviluppare questa iniziativa, però, intanto vi chiediamo gli eurobond per le infrastrutture, la gestione di quote europee del debito se proporzionali alla dimensione del prodotto di ogni Paese. Cioè, vogliamo davvero una nuova *governance* economica europea, contro il conservatorismo della Germania. Ma contro il conservatorismo della Germania, non si può andare senza mettere a posto la nostra condizione di partenza, perché non siamo credibili. Sarebbe come un noto rapinatore che vuole proporre di ridurre le pene per le rapine in banca. Non funziona. Funzionerà soltanto se noi prima rendiamo credibile, attraverso quello che ci siamo impegnati a fare - voi vi siete impegnati a fare, il Governo si è impegnato a fare - niente di più e niente di meno, il nostro impegno,

nell'attuale momento politico. È vero che all'interno dell'Unione europea, in questo momento, si stanno discutendo le regole alle quali gli Stati membri dovranno attenersi in materia di finanza pubblica. Il nome è detto chiaramente, Patto di stabilità e crescita, ma di fatto siamo di fronte alle norme di finanza pubblica. Di questo si tratta. La posizione del collega Morando è la seguente. È questa la sede per poter introdurre le norme che ci vengono richieste in sede europea?

le questioni che stanno a cuore all'Italia come, per esempio, gli eurobond per le infrastrutture, uno dei temi che il nostro Governo ha posto all'interno dell'Unione

Possiamo in questo momento, prima dell'accordo in sede di Unione europea, definire esattamente in detta sede, che è particolarmente autorevole, i parametri fissi ai quali attenerci? L'emendamento 2.4 (testo 2), che è uno dei più importanti, fissa, per esempio, il parametro di Mi chiedo se, una volta e pluriennalmente, ma addirittura senza alcun termine, e in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, si possa fissare in questo momento esattamente quel parametro, che - lo ripeto - ha natura

veicolo legislativo nel quale stabilire quali sono i parametri ai quali attenersi. Peraltro, personalmente non sono certo che un parametro possa essere fissato in maniera rigida e per un tempo indefinito senza tenere conto della mutevolezza delle condizioni economiche e finanziarie. Ovviamente viene posta una obiezione dal collega dell'opposizione, perché si riferisce all'indebitamento netto strutturale, un indebitamento cioè che tiene conto del ciclo. Ma ci troveremmo di fronte alla seguente situazione: per un verso, una percentuale fissa, lo 0,5; per altro verso, una definizione, l'indebitamento strutturale, che ha bisogno di di anno in anno di una verifica per comprendere quali sono gli effetti del ciclo economico sull'indebitamento netto strutturale, tanto che la Germania ha invece introdotto un parametro fisso nella sua Costituzione. Credo che la situazione dell'Italia necessiti di

e di un rientro del debito altrettanto significativo: su questi punti non credo ci sia differenza. Penso però che né il veicolo, antecedente alla fissazione delle grandezze all'interno dell'Unione europea, né la rigidità del numero possano, nella situazione italiana, essere introdotti. Lo sforzo che dobbiamo fare è quello di

e questo ci accomuna, senatore Morando - che non possiamo rinviare tutto al 2014 o al 2015, perché intanto

contenimento dell'indebitamento annuo che consentano all'Italia di stare bene nell'Europa e nell'euro. Ritengo - e questo non

Alla luce di ciò che, in sede UE, il nostro Governo riuscirà a ottenere, penso che si possa giungere a una più efficace sistemazione e valutazione

all'introduzione, in qualche modo, del debito privato, del risparmio privato che dir si voglia, all'interno dei parametri da valutare circa la situazione complessiva del proprio Paese. O non è quello il momento in cui, insieme,

alla riflessione del Parlamento anche questo elemento di opportunità politica, perché è giusto che, nel momento della trattativa complessiva, il Governo abbia tutte le

attenersi rigorosamente ai parametri fissati in sede europea, non credo che questo sia il momento e la sede adesso più opportuna. Esclusivamente

numerico del parametro: lo 0,5 piuttosto che lo 0,4 e lo 0,7 a me pare un elemento di rigidità che in questo momento, prima di una fissazione in sede europea, nuocerebbe all'azione complessiva del nostro Paese all'interno di quel consesso.

Senatore Viceconte, lei deve votare e stare al suo posto. **Il Senato non

gli argomenti che sono stati portati anche in ultimo contro l'approvazione di questo emendamento semplicemente non sono fondati. Dice il relatore di maggioranza: una volta che saranno stati fissati gli obiettivi di medio termine, allora avrà un senso introdurre queste regole nella legge di contabilità, o addirittura, come fanno altri Paesi, nella Costituzione, ma questi obiettivi non sono ancora stati fissati, e quindi non è giusto fare subito questa scelta. Si dà il caso - insisto, signor relatore - che questi obiettivi siano già stati fissati. fissati. Infatti nel documento dei Capi di Stato e di Governo si dice chiaramente che le regole da introdurre nella legislazione nazionale sono quelle conseguenti all'applicazione del Patto di stabilità e crescita così com'è. nel Patto di stabilità e crescita così com'è, è scritto che noi abbiamo un obiettivo di medio termine che è il pareggio di bilancio infrastrutturale essendo un Paese che non ha ancora raggiunto questo obiettivo, dobbiamo migliorare ogni anno. Ecco perché abbiamo previsto la cifra dello 0,5 per cento: non l'abbiamo scritto noi, è scritto nel Patto di stabilità e crescita. Il Paese che non ha ancora raggiunto - e noi purtroppo siamo tra questi - l'obiettivo di medio termine deve migliorare l'indebitamento strutturale dello 0,5 per cento del PIL ogni anno rispetto all'anno precedente. allora la novità? La novità non consiste né nella determinazione del parametro né nell'esistenza stessa del parametro, ma nel fatto che, nella nuova *governance* economica europea, i Capi di Governo si sono impegnati ad introdurre nella legislazione nazionale regole volte al conseguimento di questi obiettivi.

e non c'è nemmeno una determinazione quantitativa di obiettivi che non sia già stata definita in sede europea. La prova è data, se ce ne fosse bisogno, dallo stesso comunicato dei Capi di Governo dell'11 marzo, i quali dicono esplicitamente: «Il Patto» quello che qui è descritto - «sarà formalmente adottato in sede di Consiglio europeo del 24 marzo dagli Stati membri della zona euro» - e questa è una decisione presa ecco la novità che si potrebbe introdurre nei giorni 24 e 25 marzo - «dagli Stati non euro che potranno decidere di aderirvi», e lo dovranno dire il 24 e il 25 marzo. Continua il documento: «Gli Stati membri in grado di farlo dovrebbero annunciare» - e noi vogliamo mettere il Governo in grado di ottemperare a questo impegno che si è preso

assieme alla Germania e alla Francia, a dire che l'Italia, Stato fondatore dell'Unione, è in grado di precisare da subito che si sta dotando - come sta facendo la Francia e come purtroppo per noi ha già fatto la Germania, perché è arrivata di gran lunga prima di noi - delle regole necessarie per rendere più severo il Patto. Questa è la nostra proposta, e francamente non ci trova d'accordo né l'argomento relativo al fatto che la decisione sarà presa e non lo è ancora perché è dimostrato *per tabulas* che non è fondato - né quello sulla determinazione quantitativa dell'obiettivo che sarebbe imprudente fissare nella legge di contabilità. Se è imprudente fissarlo nella legge di contabilità, quanto è imprudente averlo già fissato nel 2005, quell'obiettivo quantitativo, nel Patto di stabilità e crescita europeo? Sono argomenti che a mio modesto giudizio non stanno in piedi. La verità, signor Presidente, signori della maggioranza, signori del Governo - me ne rendo conto - è questa: sapete cosa vuol dire prendere questa decisione a proposito del controllo della spesa corrente primaria, della spesa nominale? Prendere questo orientamento, a cui ci obbliga il Patto di stabilità e crescita così come definito nel 2005, significa che di qui al 2017 ogni anno dobbiamo migliorare dello 0,5 per cento l'indebitamento strutturale e significa che la spesa nominale delle amministrazioni non deve crescere rispetto all'anno precedente. È chiaro che si tratta di un obiettivo estremamente ambizioso; ma d'altra parte, se non conseguiamo questo obiettivo e perdiamo i tre anni che ci separano dal 2014 sono proprio curioso di vedere come faremo nel 2014 - per miracolo - a recuperare tutta la strada che nel frattempo non avremo percorso. Se non conseguiamo questo obiettivo, che vogliamo fare? Vogliamo uscire dall'euro? Vogliamo mettere in discussione la presenza dell'Italia nell'Unione europea? Io credo che sia un fatto di assoluta responsabilità politica che ci si propone dinnanzi per una scelta. Noi questa scelta l'abbiamo compiuta, il Governo e la maggioranza, non perché la proposta non sia tecnicamente fondata, ma perché non reggono politicamente le conseguenze di questo provvedimento, si rifiutano di adottarla.

della spesa nominale corrente e che questa potrà dilagare sul fronte dell'aumento della pressione fiscale. Questo è l'impegno che assumiamo in sede europea.

Presidente, come potrà vedere, in seconda fila ci sono due colleghi presenti e tre voti espressi.

ai nostri lavori, comunico che la lettura del calendario, con eventuale discussione, avrà luogo alle ore 18,30.

3.2 e 3.3 sono conseguenti a quello di cui abbiamo appena discusso. Se nella legge di contabilità si fosse accettato - come noi auspicavamo

L'introduzione di quella regola avrebbe infatti indotto a questi comportamenti anche senza prevedere esplicitamente tali norme. Il fatto però che l'emendamento 2.4 (testo 2) - come prevedevamo - sia stato respinto

Signor Presidente, per dimostrare ciò, invece di illustrare specificatamente gli emendamenti in questione leggerò un brevissimo passo dell'audizione del capo del Servizio studi di struttura economica e finanziaria della Banca d'Italia, Daniele Franco, audito dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica proprio in occasione della modifica della legge di contabilità al fine di renderla coerente con la nuova*governance* economica europea. Dice il dottor Franco della Banca d'Italia: «Una volta completata la realizzazione del federalismo fiscale, la regola di spesa» - ecco il punto - «potrebbe riguardare le uscite primarie delle Amministrazioni centrali e degli Enti di previdenza». La Banca d'Italia La Banca d'Italia dice, cioè: se attraverso il federalismo abbiamo iscritto in un solido patto di stabilità interno la finanza locale mettendola in una relazione coerente e positiva con la finanza dello Stato centrale, a quel punto l'introduzione di una regola di evoluzione della spesa coerente con gli obiettivi di medio termine naturalmente per lo Stato centrale ci darebbe la garanzia della realizzazione degli obiettivi di risanamento e stabilizzazione di cui stiamo parlando. cui stiamo parlando. Ho fatto parlare la Banca d'Italia, invece di illustrare l'emendamento, per la banale ragione che l'emendamento 3.2 è traduttivo, con puntualità, di quella proposta avanzata in sede di audizione non da un pericoloso esponente dell'opposizione, ma dalla Banca d'Italia. Lo stesso discorso vale per l'emendamento 3.3, che ripropone quello che diceva prima il senatore Baldassarri.

una spesa pari per quantità a quella nuova determinata dall'innovazione legislativa. Non si potrà cioè chiamare l'evoluzione della pressione fiscale ad inseguire sistematicamente, fuori programmazione, una spesa corrente che aumenta.

nelle tribune una delegazione dell'Istituto comprensivo «Don Milani» di Villanuova sul Clisi, in provincia di Brescia, a cui va il saluto dell'Aula.

superfluo in questa sede tornare sulle argomentazioni che ho già svolto. Per questo motivo, esprimo parere contrario su tutti gli

Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto per aggiungere un'osservazione particolare a proposito dell'emendamento 3.3. Quest'ultimo riguarda le modalità di copertura delle leggi che rechino oneri, cioè o determinino un minore gettito o determinino un aumento della spesa.

«mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18» della legge di contabilità. Cosa vuol dire, colleghi (perché sembra che parliamo un linguaggio per iniziati)? Vuol dire che il Governo e il Parlamento, a inizio d'anno, prendono la decisione di bilancio; nell'assumere la decisione di bilancio appostano nello stesso, nei cosiddetti fondi speciali, le risorse necessarie per realizzare quelle nuove spese che ritengono coerenti con la loro programmazione economica e finanziaria. I fondi speciali, dunque, sono il mezzo di finanziamento di leggi di spesa (che determinino oneri: possono essere anche leggi di riduzione del gettito) che sono coerenti con l'indirizzo di politica economica e di bilancio del Governo e della maggioranza. A questo proposito, signor Presidente, cosa sta accadendo? Sta accadendo quello che dice la Corte dei conti in una relazione (i colleghi ne possono prendere visione; domani pomeriggio ci sarà un convegno a cui parteciperà il presidente della Corte dei conti proprio qui al Senato in proposito). La Corte dei conti, com'è noto, ogni quattro mesi stila una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nei quattro mesi precedenti. Nella relazione sulla copertura e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi del quadrimestre maggio-agosto 2010, la Corte dei conti scrive - non dico «come risulta dal quadro riassuntivo dei mezzi di copertura - tavola 3 in allegato - anche nel periodo in esame l'incidenza delle coperture a carico dei fondi speciali è stata pressoché nulla e pertanto i nuovi oneri non rientrano in un quadro programmatorio predefinito». Ci facciamo dire, cioè, dalla Corte dei conti: guardate che fate innovazioni legislative che determinano maggiore spesa, non usate mai i fondi speciali per coprire, questo significa quindi che spendete (si rivolge a tutti, al Parlamento nel suo complesso, perché è il Parlamento che delibera) senza alcun riferimento programmatorio, in un regime di risorse scarse. Ma riflettiamoci un attimo, a questo punto! In un regime in cui le risorse pubbliche sono estremamente scarse, e quindi dovremmo farne un uso oculatissimo, ci facciamo dire dalla Corte dei conti: fate delle leggi che determinano oneri di nuova spesa, ma non le coprite mai con i fondi speciali, cioè con le risorse che avete appostato in coerenza con la vostra programmazione. Ma è possibile che la politica (la politica nel suo insieme, maggioranza, Governo e opposizione) non abbia un sussulto di dignità, e di fronte ad affermazioni così esplicite di un organo di controllo, non dica: «ma no, io torno alla buona pratica»? Le nuove spese, in capo d'anno e via via nel corso dell'anno, si coprono sui fondi speciali. Per quale motivo? Perché così dice il buon senso, così prescrive la buona programmazione economica e così prescrive la condizione di un Paese che non può permettersi più di sperperare, senza un disegno di programmazione chiaro, nemmeno un euro. Questo dice l'emendamento 3.3. Voi lo respingerete, ma state respingendo soluzioni che sono vitali per un salto di qualità nel governo della cosa pubblica in Italia e nel risanamento della finanza pubblica.

appaiono quasi come delle tecnicalità, ma contengono una precisa scelta politica rispetto alla quale il Parlamento è chiamato ad esprimersi. La scelta politica è tra un monopolio di potere come miscela di burocrazie che fanno il gioco delle tre carte sui conti pubblici oppure vincoli di trasparenza che fanno un Parlamento consapevole di quello che sta votando e delle conseguenze in termini di bilancio pubblico, in termini di andamento di spesa ed entrate e dei loro effetti sul sistema economico. Non sono tecnicalità questi emendamenti: sono la pietra portante della democrazia economica, con un Parlamento consapevole di quello che vota su ogni provvedimento di volta in volta. Abbiamo assistito in queste Aule materia di bollinatura della Ragioneria dello Stato: nel caso del Governo di centrosinistra, si tentò addirittura di assegnarne la responsabilità responsabilità ad un Sottosegretario di Stato; nel caso di un Governo di centrodestra, si è data la bollinatura su un provvedimento che fino a poche settimane

ma della pietra portante della democrazia economica e del futuro dell'equilibrio di finanza pubblica di questo Paese. Scalfire il monopolio di potere dei conti pubblici è dovere collettivo

emendamenti. Con riguardo agli emendamenti 4.1 e 4.100, di identico contenuto, dichiaro inammissibile la lettera *b)* di tali proposte, in quanto volta a disciplinare, con legge,

«In relazione a quanto previsto dal comma 1,» ‑ che questo provvedimento non modifica ‑ «i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell'attività istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti,» - attenzione: si parla dei Presidenti della Camera e del Senato nella legge vigente «adottano intese volte a promuovere le attività delle due Camere, anche in forma congiunta, nonché la collaborazione tra le rispettive strutture di supporto tecnico». Ora, Presidente, questa legge è in vigore: ne deduco che *illo tempore* i Presidenti della Camera e del Senato abbiano considerato ammissibile un testo - non importa se un emendamento

anche il testo dell'emendamento, che lascia inalterato il meccanismo delle intese tra Presidente della Camera e Presidente del Senato? Se i Presidenti non fanno le intese, non si farà alcuna integrazione, perché l'integrazione in tanto c'è in quanto ci sia l'intesa per promuoverla.

che contiene questa disposizione circa le intese tra Presidente della Camera e Presidente del Senato si dichiari inammissibile un emendamento che propone semplicemente di stabilire che, oltre alla collaborazione, queste intese possano promuovere I Presidenti di Camera e Senato sono liberissimi: fanno l'intesa per la collaborazione? Rimarrà la collaborazione. Fanno l'intesa prevedendo anche l'integrazione? Si farà pure l'integrazione. Non fanno alcuna intesa?

Sollecito pertanto i colleghi a considerare l'opportunità, se si ritiene, di respingere politicamente l'emendamento, ma di suggerire alla Presidenza di consentire lo svolgimento di un dibattito

parleremo), stanno procedendo tutti i Paesi europei, uno dopo l'altro, perché si tratta di una scelta iper-raccomandata dalla Commissione e dall'OCSE per la trasparenza dei conti pubblici, che - come sapete - per un Paese molto indebitato

I termini sono stati posti in modo assolutamente preciso dal collega Morando. Io le chiedo, a nome del Gruppo, formalmente di riesaminare questa decisione di inammissibilità. Sarebbe un precedente gravissimo

Si è posto in passato il tema della non possibilità per il legislatore di intervenire sulle materie riservate ai Presidenti delle Camere. Credo che i colleghi ricorderanno bene che questo tema si pose, ad esempio, a proposito della possibilità o meno di imporre alle Camere

specifico, del Presidente del Senato e dei Presidenti delle Camere, ma può stabilire un percorso, un obiettivo dentro il quale si esercitano le prerogative dei Presidenti delle Camere. Ed è esattamente ciò che afferma sia l'articolo 4 della legge di contabilità

Peraltro, signor Presidente, ricordo a lei e ai colleghi che proposte emendative di questo tipo noi le abbiamo formulate in numerosi altri provvedimenti, anche in occasione - credo di ricordare - dell'esame della legge di stabilità o dell'esame di provvedimenti finanziari in quest'Aula, e mai era stata adottata una decisione di inammissibilità come quella che oggi ci viene prospettata. Quindi, non ci accontentiamo, signor Presidente,

i Presidenti delle Camere, nella loro totale autonomia, possono fare intese volte a promuovere l'integrazione. Quindi, francamente non capisco, in lingua italiana, oltre la legge vigente, quale sia il punto di lesione dell'autonomia delle due Camere.

alla possibilità del Senato di entrare nel merito di un argomento che era stato anche oggetto di modifiche rispetto alla legislazione vigente da parte della Camera. Non possiamo però accogliere la proposta

Stiamo parlando di come il Parlamento intende organizzarsi per affrontare due grandi rivoluzioni in corso. prima rivoluzione certa riguarda il fatto che si modifica profondamente il quadro europeo di coordinamento della finanza pubblica. Il Governo tende a minimizzare queste scadenze, ma chiunque legga i documenti che sono stati sottoscritti, come ricordato dal senatore Morando, sa che si tratta di una vera e propria rivoluzione. La seconda rivoluzione, che rischia magari di essere più annunciata che realizzata, riguarda il federalismo. Comunque sia, pur con le incertezze e le contraddizioni con cui si sta dando attuazione alla delega, non c'è dubbio che si modificherà profondamente il sistema della finanza centrale e il suo rapporto con il sistema della finanza regionale e locale. Abbiamo quindi di fronte due autentiche rivoluzioni, che noi vogliamo prendere sul serio. Come si può pensare che tutto resti uguale se si innovano così profondamente le procedure di bilancio ed i rapporti tra i diversi livelli di decisione di bilancio? Noi manteniamo le stesse strutture del secolo scorso, anzi, di due secoli fa, per alcuni aspetti; com'è possibile non sentire l'esigenza di di cogliere questa sfida anche attraverso un ammodernamento delle nostre strutture? È infatti in corso un duplice spostamento delle procedure, dai Governi nazionali alla sede comunitaria, finalmente ci si sta rendendo conto, sotto la pressione della crisi, che la moneta comune richiede anche di incominciare ad approntare una comune gestione finanziaria, almeno coordinata sui grandi flussi e sui grandi indirizzi. è poi uno spostamento di potere reale dai Parlamenti ai Governi, reso necessario dalla complessità delle decisioni che si devono assumere.

e un controllo pubblico all'interno di un regime parlamentare e far sì che questa occasione non si traduca in un impoverimento delle funzioni del Parlamento ma in un arricchimento e in un ammodernamento? È evidente a tutti che questo nuovo quadro sottolinea alcuni aspetti. Il primo è quello della necessità di un'autorità indipendente nella valutazione della situazione della finanza pubblica: tutta la vicenda della crisi e dei rischi di stress della finanza pubblica dimostra che c'è bisogno di una struttura di questo tipo. il problema del controllo democratico della conduzione della finanza pubblica in un sistema molto più complesso e multilivello. il problema di concentrarsi con più attenzione alla fase *ex* *post*. Noi ci concentriamo molto sulla fase *ex* *ante,* nel valutare le coperture più o meno realistiche dei provvedimenti, in sintonia con l'articolo 81 della Costituzione, ma molto poco conosciamo della fase *ex post*. Conoscere bene anche la fase in essere una lotta autentica agli sprechi e anche affrontare il grande tema della lotta alla corruzione, perché con la trasparenza si combattono i fenomeni degenerativi; significa inoltre istituzioni più vicine al cittadino, perché in grado di motivare le decisioni e farne conoscere la natura profonda. Tutto questo non è un grande problema? Non si tratta di una tecnica organizzativa, ma di una questione che attiene all'efficacia delle procedure di bilancio e alla qualità del processo democratico. dunque che ci sarebbero per questi motivi piene ragioni di approvare questo nostro emendamento. Insisteremo comunque anche nel futuro, per i motivi che ho espresso brevemente, ricordando tuttavia, signor Presidente, si può essere contrari a questo emendamento ma, secondo me, questa contrarietà denota miopia e anche poco affetto all'istituzione parlamentare. C'è però una legislazione vigente

ogni volta ci è stato detto che sarebbe stato opportuno rinviare la discussione ad altro provvedimento più consono e coerente. Questa motivazione francamente non è accettabile, almeno da parte mia,

di un punto cruciale per la democrazia e per il ruolo del Parlamento: mi riferisco all'istituzione di un'autorità di controllo della finanza pubblica, che è fondamentale per dare certezza e trasparenza ai conti pubblici. Per un Paese con un alto debito pubblico come l'Italia, questa certezza e questa trasparenza nel tempo, nei confronti dei mercati finanziari, può valere una riduzione dello *spread* sui *Bund* tedeschi tedeschi forse di parecchi punti base. Quindi, è un elemento anche quantificabile sul piano economico. Come ho detto in precedenza, le vicende di questi ultimi anni dimostrano la crucialità e l'importanza dell'istituzione di una autorità di finanza pubblica, proprio in base agli esempi che tutti abbiamo vissuto in questa Aula, sia nel ruolo di maggioranza che di opposizione, nelle alterne vicende dei Governi che si sono succeduti. Ricordo che lasciare la situazione attuale significa lasciare le condizioni di finanza pubblica nella pressoché totale arbitrarietà di alcune burocrazie, di affidarle a un'autorità indipendente. Da questo punto di vista, l'esempio più evidente è quello che abbiamo vissuto poche settimane fa:

la necessità di una copertura per una caduta del gettito stimata in 2,8 miliardi di euro; improvvisamente, quello stesso provvedimento, inserito nel federalismo municipale, ha avuto una stima della Ragioneria generale dello Stato di maggiore gettito

che per trent'anni, ogni anno, i Governi che si sono succeduti hanno proposto al Parlamento manovre di tagli di spesa e di aumenti di tasse. tasse. Qui giace il grande mistero della finanza pubblica italiana: se dopo trent'anni di manovre di tagli di spesa e di aumenti di tasse ci ritroviamo con il terzo debito pubblico del mondo, si tratta di un miracolo. È evidente allora che i tagli di spesa non erano tali e gli aumenti di tasse in parte erano veri, in parte erano lotta all'evasione, che è *ex post* e non è mai stata misurata. Il risultato è stato quello di ritrovarci con questo macigno di debito pubblico. Se vogliamo sul serio affrontare, come è urgente e necessario, il problema del debito, dobbiamo in primo luogo dare chiarezza e trasparenza a tutta la finanza pubblica, problema che diventa più complicato proprio con l'attuazione del federalismo fiscale e quindi della responsabilità dei vari bilanci che fanno parte del perimetro della pubblica amministrazione. Quindi, invito il Governo e il relatore a riflettere ulteriormente su quel parere contrario, perché senza una autorità indipendente che riferisca al Parlamento, e magari anche al Governo, i dati certi sulla finanza pubblica, correremmo i rischi che sono diventati la triste realtà di questi trent'anni, nei quali il Parlamento votava leggi finanziarie che apparentemente apparentemente tagliavano il deficit e rallentavano il debito, ma che di fatto aumentavano il deficit nascondendolo, e aumentavano il debito pubblico. Questa è la realtà dell'emendamento. Credo che questa sia la quarta o quinta volta, almeno per quello che mi riguarda, viene sottoposto all'attenzione dell'Aula e dei colleghi, e credo che altrettanto abbia fatto, nel corso degli anni, il collega Morando.

Presidente, l'Aula ha appena respinto un importante emendamento che, grazie alla modifica del parere di ammissibilità, era stato posto in votazione. Il nostro Gruppo, in in conseguenza di tale bocciatura, richiama l'attenzione sull'emendamento 4.0.2. Con tale emendamento, signor Presidente, si chiede l'istituzione di un'autorità indipendente per la trasparenza dei conti pubblici. È bene fare qualche precisazione in proposito, in modo che i colleghi siano in grado di assumere le necessarie determinazioni in ordine al voto. Le autorità fiscali, signor Presidente, dovrebbero contribuire a ridurre il noto *deficit bias*, ossia la tendenza dei disavanzi pubblici ad aumentare e quella del debito ad accumularsi. Considerazioni di opportunismo intergenerazionale possono spesso indurre il decisore politico ad adottare politiche che favoriscano gli elettori presenti rispetto a quelli futuri, ad esempio intraprendendo programmi di aumento della spesa o di riduzione delle imposte non coerenti con una sostenibilità di medio periodo, per ottenere il consenso necessario alla loro rielezione: è il famoso ciclo elettorale. Una seconda modalità di *deficit bias* può essere dovuta a problemi di *common pool*, in quanto vi può essere la tendenza ad incrementare programmi di spesa e riduzione di imposte che favoriscano uno specifico gruppo d'interesse, senza che questo sostenga l'onere integrale del finanziamento. L'ultimo problema è quello del *time inconsistency*, ossia delle situazioni nelle quali il Governo, il decisore politico, si impegna *ex ante* ad adottare determinate misure di *policy*, ma poi *ex post* non rispetta gli obiettivi in quanto considerazioni di altra natura prendono il sopravvento. Nel caso italiano, colleghi, le problematiche che più ci convincono a propendere per la costituzione di un *fiscal council* sono essenzialmente due: la prima è la sfida del consolidamento; la seconda è l'attuazione del federalismo fiscale, tanto caro a tutti (quindi vi pregherei di ragionarci su), con i conseguenti problemi di *common pool* e di asimmetria informativa. Sempre nel nostro caso italiano, signor Presidente, è auspicabile l'introduzione di un'istituzione che svolga funzioni legate alla trasparenza e alla disponibilità di informazioni. Spesso viene sottolineata l'importanza di rompere il cosiddetto monopolio informativo, oggi totalmente nelle mani dell'Esecutivo e, per esso, del Ministro dell'economia.

un ambito forse troppo suscettibile di contestazione politica, aspetto che quindi indebolirebbe questa nuova istituzione. In realtà, signor Presidente, non solo nel dibattito in Commissione, dove quest'anno, rispetto a due anni fa (quando approvammo il disegno di legge di riforma della disciplina di bilancio), c'è stata molta più apertura all'idea di un'*authority* indipendente, ma anche in generale, sia a livello accademico che in gran parte del mondo politico (che si differenzia fra gli interventi in Aula e quelli fuori dalle Aule parlamentari dove si vota), vi è un generale consenso sull'importanza di creare autorità fiscali indipendenti dal potere politico, come diretta conseguenza di quanto detto in precedenza a proposito di quel *deficit* spesso collegato a distorsioni del sistema politico. Tra gli elementi fondamentali che sono utili a garantire l'indipendenza di questa istituzione è opportuno segnalarne alcuni, affinché rimangano agli atti. *In primis*, vi è il divieto per il Governo di interferire con l'attività dell'autorità fiscale e per l'istituzione di ricevere istruzioni da parte dell'Esecutivo. In seconda battuta, gli incarichi dei rappresentanti dell'autorità fiscale devono durare più di una legislatura ma non devono essere rinnovabili. limiti severi per il Governo alla revoca della nomina dei membri che compongono il *board* dell'autorità fiscale. Le procedure di nomina devono privilegiare requisiti tecnici piuttosto che considerazioni di carattere puramente politico. I membri del *board* dell'autorità dovrebbero essere selezionati, in misura variabile, tra accademici, analisti del settore finanziario ed esperti di finanza pubblica che abbiano lavorato all'interno della pubblica amministrazione. I criteri di finanziamento dovrebbero garantire la continuità dell'attività e, quindi, non dovrebbero essere sottoponibili a tagli. Signor Presidente, l'analisi delle esperienze internazionali, spesso citate negli interventi che mi hanno preceduto, svolta per quanto ci riguarda dal prezioso Servizio del bilancio del Senato, che continuo a ringraziare pubblicamente, dimostra dimostra che l'indipendenza dipende più dalla volontà di riconoscere tale funzione da parte di tutto il sistema politico che non dalle caratteristiche istituzionali scelte per il funzionamento dell'organismo stesso. La competenza delle persone che ci lavorano e che lo dirigono dovrebbe essere indiscussa (aspetto quest'ultimo, che è particolarmente rilevante soprattutto nel periodo di *start up*, cioè di costituzione della reputazione di questo organismo).

che l'incardinamento presso il Parlamento è più difficile da realizzare: basti pensare all'emendamento appena bocciato che richiamava una norma della legge n. 196 del 2009 che prevedeva che avvenisse con atti interni, le famose intese (questa la formula usata nella legge n. 196) che, pur previste da una legge di riforma (la legge di bilancio del 2009), non sono mai state adottate

avrebbe una maggior difficoltà di realizzazione, ma sarebbe anche più difficile da smantellare, cosa che invece servirebbe molto a questo Parlamento. Per questo motivo invito i colleghi a valutare bene l'opportunità - vedo che c'è un emendamento molto simile

Presidente, noi voteremo a favore dell'emendamento 4.0.100 (testo 2), presentato dal senatore Baldassarri e da altri colleghi. Lo faremo malgrado - credo sia risultato chiaro nella discussione che ha preceduto la votazione di questo emendamento - noi si preferisca tra le possibili soluzioni per la costruzione in Italia di autorità indipendenti per il controllo e la valutazione degli andamenti di finanza pubblica la soluzione dell'incardinamento della costruzione di questo *fiscal council*, come viene chiamato usando un'altra lingua, presso il Parlamento e non fuori. Perché voteremo dunque a favore di un emendamento che propone la costruzione di una autorità esterna? Perché dobbiamo purtroppo constatare quella pervicace opposizione alla soluzione di incardinamento presso il Parlamento del nuovo Servizio del bilancio del Parlamento italiano nel suo complesso che ancora una volta si è manifestata questa sera. colleghi, io credo di essere facile profeta. Sappiamo che sia l'OCSE sia la Commissione europea stanno praticamente ad ogni occasione raccomandando agli Stati (nel caso dell'OCSE agli Stati membri dell'OCSE, nel caso della Commissione europea agli Stati membri dell'Unione) di dotarsi di istituzioni per l'analisi dei conti pubblici e per le valutazioni economiche relativamente indipendenti. Perché? Perchè, nel momento in cui si definisce la nuova *governance* economica europea e si definiscono obiettivi di lungo periodo (l'obiettivo di medio termine è a 10 anni nella nuova *governance* economica europea). È chiaro allora che l'affidabilità delle valutazioni previsionali dei tendenziali non può derivare solo dalla analisi delle istituzioni costruite in seno ai Governi: ci deve essere una autorità indipendente che abbia una relazione fortissima, in termini di possibilità di utilizzare gli stessi dati e le stesse informazioni, con gli uffici del Governo, ma abbia un carattere di relativa autonomia. Faccio una previsione: o noi ci decidiamo a costruire il Servizio del bilancio del Parlamento europeo attivando le intese previste tra Camera e Senato dall'articolo 4 della legge di contabilità, o nei prossimi mesi sarà il Governo, prendendo atto dell'inattività del Parlamento sul punto, a procedere alla costruzione di una autorità indipendente. Vogliamo questa soluzione? Continuiamo a comportarci come abbiamo fatto poco fa nella votazione dell'emendamento favorevole alla costruzione di un Servizio del bilancio del Parlamento italiano. Siccome quell'emendamento è stato respinto io, che pure sono fermamente contrario alla costruzione di questa autorità fuori dal Parlamento (perché sono per l'applicazione in Italia del modello del *Congressional Budget Office* americano - la più

di fronte alla negazione di tale possibilità non posso far altro che votare a favore anche dell'emendamento che propone l'autorità esterna. un piccolo episodio che dimostra qual'è la qualità della politica se c'è l'Ufficio del bilancio del Parlamento oppure se non c'è. Nel marzo 2009 il CBO, *Congressional Budget Office* americano, fa uscire uno studio clamoroso in cui dice che dei 700 miliardi di dollari di spesa previsti per l'attuazione del cosiddetto piano Paulson, il piano cioè di intervento sulla crisi fatto proprio sostanzialmente dall'amministrazione

Il giorno dopo tutti i grandi giornali della destra americana, del partito repubblicano, escono più o meno con un titolo così: lo conferma il CBO, con Obama gli Stati Uniti sono uno Stato socialista. La replica della sinistra - dei *liberal*, dei *democrat* americani - è durissima contro questo tipo di battaglia, ma nessuno, né da una parte né dall'altra, nel corso di quella discussione ha messo in discussione la validità dello studio. I democratici si sono difesi negando che stesse prevalendo un orientamento socialista e anzi sottolineando che era stata l'amministrazione della destra a far emergere quel piano e ad approvarne le prime scelte; i repubblicani hanno insistito sulla loro interpretazione; ma nessuno ha messo in discussione i dati, i dati, malgrado il putiferio. Perché scoppiò negli Stati Uniti un vero e proprio putiferio a causa di quello studio, e nel giugno dello stesso anno il CBO, imperterrito, fece uscire uno studio nel quale diceva: sono stati già spesi 300 miliardi di dollari; di questi 300 miliardi di dollari ne sono stati recuperati, come noi vi avevamo detto, poco più di 150, e ribadiva papale papale il suo studio precedente. Ora, se noi fossimo in un Paese nel quale c'è qualcosa di simile, in Italia, noi discuteremmo sulle soluzioni di destra o di sinistra del problema che nasce dalla valutazione della realtà, ma non staremmo a litigare sulla descrizione con i numeri dei dati di finanza pubblica. Sarebbe un passo in avanti per la politica italiana formidabile. Io ho una grande ammirazione per quegli Stati che sono in grado di realizzare intese tra destra e sinistra per migliorare la base del loro confronto e del loro conflitto. Fermo restando che il confronto e il conflitto negli Stati Uniti d'America, anche grazie all'esistenza del CBO, è più duro nel merito di quello che non sia in Italia, ma non riguarda la sparatoria sul pianista, sul conducente, su quello che ha la sola responsabilità di analizzare con un minimo di obiettività e con indiscussa autorevolezza i dati. Potete continuare, colleghi della maggioranza, a dire di no a questa soluzione, ma prima o dopo vi troverete costretti a scegliere, per non avere mangiato questa minestra, di saltare dalla finestra, cioè a creare in Italia un'autorità fuori dal Parlamento che non sarà mio giudizio, per come è organizzato il sistema politico italiano, di fornire tutto quel contributo e quel servizio di merito che potrebbe essere fornito dalla costruzione di un grande ufficio del bilancio presso il Parlamento italiano. Prima o dopo ci arriveremo; noi non intendiamo desistere. Questa è una battaglia sacrosanta: non è una battaglia di destra, non è una battaglia di sinistra, è una battaglia delle persone ragionevoli e prima o dopo la vinceremo, contro i conservatori di tutti i campi.

L'ordine del giorno della seduta odierna prevede il seguito della discussione del disegno di legge relativo alle modifiche alla legge di contabilità e finanza pubblica. Nella seduta antimeridiana di domani sarà esaminato il decreto-legge recante disposizioni sulla festa nazionale del 17 marzo 2011, per il quale si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi. Nella seduta pomeridiana di domani - per la quale non è fissato l'orario di chiusura - sono previste comunicazioni del Governo sulla crisi libica. Seguirà un dibattito che potrà concludersi con la votazione di strumenti di indirizzo, ove presentati. Su questo punto la Conferenza si è pronunciata a maggioranza. Nella seduta antimeridiana di giovedì 24 marzo saranno discusse mozioni sulle energie rinnovabili. L'esame del disegno di legge recante modifiche al codice di procedura penale a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, già previsto per la settimana corrente, è stato differito alla prossima settimana, con l'intesa che avrà luogo anche ove non concluso dalla Commissione. Il calendario della prossima settimana prevede inoltre l'esame del disegno di legge sulla disciplina della rappresentanza istituzionale locale degli italiani residenti all'estero, ratifiche di accordi internazionali, il seguito dell'esame dei disegni di legge sulle squadre investigative comuni sovranazionali, nonché la discussione della mozione Micheloni sulla razionalizzazione della rete diplomatico-consolare italiana. **Programma dei lavori

Ricavo dalla lettura del suo *speech* che la richiesta che è stata avanzata dal Gruppo del Partito Democratico oggi in Conferenza dei Capigruppo, e cioè che a riferire in quest'Aula e ad assistere alla discussione che quest'Aula dovrà sostenere

Le dico che noi non siamo in condizione di votare il calendario se non sappiamo che cosa stiamo votando. Poiché oggi in Conferenza dei Capigruppo la richiesta del Gruppo del Partito Democratico è stata che venisse a riferire sulla Libia il presidente Berlusconi e non uno

Il mio Gruppo ha sospeso ogni determinazione attendendo che da parte del Ministro per i rapporti con il Parlamento venisse la conferma o meno della presenza del presidente Berlusconi, annunciando che, qualora il presidente Berlusconi non potesse essere presente domani in Aula, il nostro Gruppo avrebbe avanzato altre ipotesi di calendario da porre in votazione e non avrebbe votato il calendario che è stato oggetto del suo *speech*. Presidente Finocchiaro, mi comunicano che alla Presidenza è arrivata la notizia che verranno i ministri Frattini e La Russa. Presidente, come avrà capito, il nostro Gruppo, che si era già attivato con una lettera a firma mia e del presidente Franceschini per chiedere che la questione che riguarda la nostra partecipazione alla missione in Libia venisse discussa in Aula e non soltanto in soltanto in Commissione, è fermo sul punto che a questa valutazione del Parlamento e a questa discussione, che sarà conclusa - come è normale che sia - da una risoluzione, sia presente il Presidente del Consiglio. Lo richiede non soltanto la delicatezza e la qualità della questione ma anche - me lo lasci dire una incertezza che si fa di ora in ora più vistosa e che ha molto a che fare con la credibilità del nostro Paese, con la qualità della nostra presenza sullo scenario internazionale, fra i Governi che partecipano

La natura dell'intervento che sto facendo mi obbliga ad essere breve, ma non posso sottacere il fatto che abbiamo sentito un Ministro, il ministro Bossi, che, parlando del Ministro della difesa, che aveva espresso alcune valutazioni sulla partecipazione dell'Italia a questa missione, appunto del ministro La Russa che «parla a vanvera», mentre ieri sera, in diretta TV ,il vice ministro Castelli e il ministro La Russa hanno avuto uno scontro pubblico esattamente sulle modalità di partecipazione, sulle ragioni che hanno motivato la decisione, sui tempi della decisione e sulla stessa natura e validità della decisione di partecipare alla missione in Libia. Forti come siamo dell'atteggiamento responsabile delle opposizioni, che abbiamo manifestato con nettezza e coerenza dal primo momento e peraltro in piena aderenza con la posizione che è stata più volte espressa e ripetuta dal Presidente della Repubblica, noi chiediamo che sia il Presidente del Consiglio

nello scenario delle forze dei Paesi che partecipano alla missione in Libia. Non dovrebbe essercene bisogno: il Governo italiano, nella persona del Presidente del Consiglio, ha partecipato al vertice di Parigi e, prima, ad una preriunione con gli Stati Uniti, con la Gran Bretagna e con la Francia. Il nostro Paese ha aderito alla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, eppure ogni giorno, dall'interno della maggioranza e da una forza che costituisce un pezzo importante, definitivo di questa maggioranza e che conta moltissimi Ministri nella compagine governativa,

di poterlo dire - dell'onore e della credibilità dell'Italia sullo scenario internazionale, e in questa vicenda in particolare. Questa non è roba che si può nascondere sotto al tappeto, perché la divaricazione interna alla maggioranza che si tende a non mostrare purtroppo purtroppo si mostra con ogni evidenza e in sedi che non sono quelle proprie, quelle istituzionali, dove dovremmo misurarci tutti (noi lo faremo con il nostro senso di responsabilità) su tale questione. Io, pertanto, avanzo due proposte alternative alla sua proposta di calendario. La prima è che il presidente Berlusconi

Berlusconi venga dinnanzi al Parlamento. Lo ha fatto Zapatero, lo ha fatto Fillon, lo sta facendo Obama, lo ha fatto Cameron. Non vedo ragione alcuna perché su questo tema, e di fronte ad un atteggiamento delle opposizioni coerente e responsabile, il Presidente del Consiglio non debba onorare non il Parlamento, ma la funzione che esercita.

che definisco demagogiche. In quest'Aula ce lo ricordiamo tutti, presumo anche all'interno del vostro Gruppo del Partito Democratico: quando

Colleghi, al Governo. Questa è la realtà, non ho detto nessuna bugia: i nostri aerei bombardavano la Serbia, senza che il Parlamento lo sapesse. Lo abbiamo letto sui giornali, lo ripeto, senza che nemmeno le Commissioni fossero state

Questa è la realtà, parlate con i pochi cittadini che ancora vi votano, chiedete quali sono i problemi del Paese, le paure che hanno nei confronti di questo intervento. L'altro aspetto importante che porteremo avanti è quello di tutelare i contratti economici che abbiamo fatto con il Governo della Libia. Le risorse energetiche sono importanti e vogliamo evitare in tutti i modi l'aumento delle bollette dell'energia elettrica e del gas per i nostri cittadini. *(Vivaci proteste dal Gruppo PD)*. Questo possiamo fare tutti insieme in Parlamento...

Ora, signor Presidente, di proseguire nel dibattito parlamentare con lo stesso spirito unitario che ha contraddistinto il comportamento dei Gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione appena qualche giorno fa, esattamente venerdì scorso,

che ha dato mandato all'Esecutivo di svolgere un determinato ruolo nell'ambito di questa iniziativa di attuazione della risoluzione n. 1973 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Non credo che questo clima debba essere sprecato, però è evidente che il dibattito di questi giorni non ha aiutato. Ora non è nostro interesse capire

dalla circostanza di meglio organizzare la missione internazionale, ciò sarebbe oggettivamente comprensibile; qualora invece dovesse nascere dall'esigenza di cambiare

dell'operato di Gheddafi o della necessità di tenerlo lì, in questa condizione, per salvaguardare presunti interessi nazionali (che non vengono invece tutelati dalla permanenza in quei

diversa rispetto a quella che abbiamo approvato pochi giorni fa tutti insieme in Commissione, è chiaro che questo può obiettivamente rappresentare un problema

Presidente, colleghi, anche il Gruppo dell'Italia dei Valori si allinea alla richiesta

Nessuno di noi, e certamente nessuno dei colleghi della maggioranza, può nascondere la delicatezza del caso che è scoppiato qualche giorno fa e che va complicandosi di ora in ora.

risoluzione, una mozione o comunque un documento, con cui si confronterà con la maggioranza. Sembrerebbe che il presidente Bricolo si sia defilato con il suo Gruppo rispetto alla posizione del PdL e quindi dei due Ministri che domani dovranno venire a riferire. Per questo è importante che venga il Presidente del Consiglio, perché non può dire che è addolorato per la posizione difficile che vive il presidente

del Governo italiano, al punto che dal baciamano si è passati ai bombardamenti, e ci dia una spiegazione puntuale e reale che non ci possono fornire i due Ministri. Il Presidente del Consiglio ha infatti un ruolo particolare, riconosciutogli anche dalla Costituzione, e rappresenta la sintesi di tutto l'organo collegiale che egli presiede. Quindi, per tranquillità

Presidente, non entrerò nel merito della discussione perché lo faremo domani. Molte cose si potrebbero dire, ma mi sembra che impropriamente alcuni colleghi siano entrati nel merito della vicenda. vicenda. Ciò che è stato detto sui precedenti, non esaltanti per i Governi dell'epoca, del Kosovo e di altre vicende, che videro prima le iniziative militari e poi le informazioni al Parlamento, lo ricorderemo in altre occasioni.

che comporterà anche delle votazioni che mostreranno come la maggioranza ha una posizione chiara e coesa rispetto alle determinazioni dell'ONU e alla difesa dei nostri interessi strategici, economici e di sicurezza nell'area del Mediterraneo. Di questo discuteremo il voto dimostrerà che non c'è alcuna fibrillazione nella maggioranza: anzi, vedremo se ci saranno fibrillazioni nelle minoranze o se, come auspichiamo, sarà possibile una convergenza di posizioni, visto il rilievo degli impegni cui l'Italia è chiamata nel contesto internazionale e in particolare

presidente Berlusconi nel corso di questa crisi avrà modo di dialogare e discutere con il Parlamento, perché questo Governo e questa maggioranza hanno intenzione di tenere un rapporto costruttivo e trasparente con il Parlamento, a differenza di quanto avvenne in occasioni precedenti. Voteremo pertanto a favore della proposta di calendario sottoposta all'Aula Presidente, lei ha ovviamente invitato tutti noi a rientrare nei contenuti della discussione relativa al calendario. Quindi, per questa ragione le le annuncio che il Gruppo Misto, in tutte le sue componenti, voterà contro questa proposta di calendario se venisse confermata la non presenza del Capo del Governo al dibattito di domani. perché, per tante buone ragioni sostenute dai colleghi, ci sembra che la vicenda nella sua drammaticità e complessità richiami in modo inderogabile la responsabilità personale e politica del Presidente del Consiglio. Non riteniamo che possano bastare né esternazioni più o meno estemporanee rese agli organi di stampa, né sfoghi, né valutazioni di ordine personale e affettivo rispetto al leader libico. Pensiamo invece che occorra assumere responsabilmente di fronte al Parlamento

ma vogliono collaborare a definire una posizione unitaria nell'interesse del Paese. Ma, perché vi sia tale posizione, occorre che il Capo del Governo venga in Parlamento ad esprimere in modo solenne la linea definitiva del nostro Paese in questa crisi drammatica.

Ma proprio questa importanza e questa straordinarietà consigliano anche di stabilire insieme, nella ricerca di quel che unisce e che deve unire in un frangente così importante, dove è in gioco non un Governo, ma l'interesse nazionale, che è qualcosa di più: qualcosa di più: una sorta di percorso nel confronto tra Governo e Parlamento a partire dall'intervento di domani del Ministro degli esteri, o di chi per lui. Ciò, nella consapevolezza che l'intervento del Presidente del Consiglio si può rendere indispensabile man mano che evolva la situazione, e che forse non è del tutto responsabile determinare fin da subito una posizione a quel livello di responsabilità, perché ci troviamo in una situazione in continua evoluzione, che consiglia una *road map* nel rapporto tra Parlamento e Governo anziché una scelta verso una direzione immediata. Questo mi sembra la posizione da tenere, e per questa ragione credo sia opportuno votare il calendario, con questo auspicio, con questo obiettivo e con queste indicazioni.

alla prossima settimana.

purtroppo però non è ancora arrivata. Il tema dell'interrogazione riguarda il sovraffollamento del carcere di Marassi. Anche ieri mattina è avvenuta una rissa tra detenuti tunisini e albanesi che ha coinvolto 50 detenuti, ha provocato 10 feriti, tra cui uno sfregiato in modo grave.

rivolto al Ministro dell'economia e delle finanze per intervenire in merito a quanto successo a Pesaro. La Guardia di finanza, a seguito di una verifica, ha contestato alla società Croce Italia Marche srl la mancata applicazione dell'IVA relativa alle fatture emesse per i trasporti effettuati su disposizione di alcuni enti. Si tratta di un discorso particolarmente complicato e complesso, tra l'altro riguardante soltanto la Regione Marche per una interpretazione che non trova riscontro in alcuna Regione d'Italia. Costituisce una inspiegabile discriminazione e una pesante penalizzazione finanziaria della Regione stessa, la quale si trova a dover corrispondere una imposta sul servizio trasporto malati ed infermi, il cui ammontare rende più oneroso il costo del servizio, con una conseguente sottrazione di risorse finanziarie da destinare all'erogazione ad altri servizi sanitari. Pertanto, chiediamo al Ministro di rispondere in merito ad una discriminazione palese di questa Regione rispetto a tutte le altre. altre. È necessario un chiarimento rispetto agli accertamenti effettuati, che non tengono assolutamente conto della risoluzione del 16 giugno 2006, n. 83, della Direzione centrale normativa e contenziosa della Agenzia delle entrate.

Un fenomeno molto particolare che ha interessato il nostro Paese vede la concomitanza di un intervento da parte di alcune realtà a livello internazionale che hanno fatto scempio del territorio, consumandolo in maniera indiscriminata per potersi garantire una cospicua rendita che invece pesa sulle spalle dei contribuenti e di tutti i cittadini. Il Ministero Il Ministero ha frenato e ha fornito un'interpretazione rispetto alla questione delle fonti di energia rinnovabili. Attendiamo che ci sia il nuovo decreto da parte del Governo, ma nel frattempo c'è una situazione estremamente pericolosa e delicata, perché, di fronte al consumo del territorio